Grazie a tutti.

Grazie

recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, è convertito in legge

Signor Presidente, il pochissimo tempo a disposizione per le Commissioni 1a e 2a riunite per esaminare il provvedimento non ci ha consentito nemmeno di concludere

credo di interpretare il sentimento unanime della mia Commissione e anche quello dei componenti della 2a Commissione nel rappresentare il disagio per non aver potuto adempiere al mandato parlamentare, al nostro lavoro e alla nostra funzione nell'esaminare e votare questo provvedimento. Non è certo la prima volta che accade. Abbiamo assistito anche nelle scorse legislature a questa prassi. Ricordo addirittura un caso in cui fui costretto, insieme al mio Gruppo, a votare una legge finanziaria che ci era stata consegnata quarantacinque Quindi certamente non è il primo caso che abbiamo di fronte. Tuttavia è una prassi sulla quale credo che quest'Aula e il Parlamento intero debbano riflettere attentamente, da ambo le parti. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Balboni, il disegno di legge n. 897, non essendosi concluso l'esame in Commissione,

Presidente, intervengo sull'ordine dei nostri lavori su questo particolare provvedimento. Vorrei concordare con le cose che ha detto il presidente Balboni e stigmatizzare il fatto che che questo ramo del Parlamento si troverà ad approvare la conversione di un decreto-legge delicatissimo, in materia tra l'altro penale, contenente norme addirittura retroattive, in un tempo *record*. Infatti abbiamo incardinato il provvedimento ieri, signor Presidente, e abbiamo ricevuto il fascicolo degli emendamenti all'apertura della seduta della Commissione. Va detto che questo ramo del Parlamento non ha esaminato questo provvedimento non per cattiva volontà o perché i Regolamenti parlamentari sono farraginosi; questo ramo del Parlamento non ha potuto esaminare il provvedimento perché ci è stato trasmesso dalla Camera il 29 settembre. Questo è un decreto-legge in data 10 agosto e quindi vuol dire che scade il 9 ottobre; noi praticamente non abbiamo potuto lavorarci. Ora, il presidente Balboni ha fatto riferimento a un disegno di legge di bilancio che era stato consegnato al Parlamento pochi minuti prima dell'approvazione al Senato. Voglio ricordare che in quell'occasione il Gruppo Partito Democratico, che era il partito al quale tra l'altro appartenevo, presentò un ricorso alla Corte costituzionale per un conflitto di poteri, lamentando proprio il fatto che la funzione parlamentare legislativa fosse stata violata. In quell'occasione, la Corte costituzionale ebbe a pronunciarsi sulla materia (quindi abbiamo un precedente), riconoscendo addirittura in capo a ciascuno di noi, signor Presidente, cioè in capo a ciascun parlamentare, la possibilità di adire la Corte ove mai ritenesse che le sue prerogative di legislatore fossero state violate. Quella volta a cui si riferisce il presidente Balboni, la Consulta non si era ancora pronunciata; ma questa volta lo ha fatto e ciò vuol dire che questa pratica deve assolutamente cessare. Noi ci troviamo in una sorta di monocameralismo alternato, nel senso che ogni ramo del Parlamento sostanzialmente guarda metà dei provvedimenti legislativi. Questa è una violazione palese della Carta costituzionale che non può essere sopportata. Aggiungo un'ultima questione: il problema è che noi siamo arrivati così tardi

che ormai si sta sfiorando una prassi che in qualche modo esautora le Camere, che possono solo guardare i documenti che arrivano dal Governo.

che ha visto un decreto-legge uscire dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto e una lettura fatta in ventiquattro ore, a metà settembre, in un solo ramo del Parlamento. Se è vero, come è vero, quello che anche il senatore Balboni ha ricordato e cioè che ormai da molto tempo le Camere sono spesso mere ratificatrici di provvedimenti d'urgenza dei Governi che si sono succeduti negli ultimi anni, è anche vero che la forza di maggioranza relativa di questo Parlamento ci ha fatto una battaglia feroce nella scorsa legislatura, promettendo che ciò non sarebbe più accaduto quando avrebbero governato loro e oggi, invece, il Governo Meloni sta battendo ogni *record* di decretazione d'urgenza e di fiducia nelle Aule parlamentari *(Applausi)* con decreti tutti *omnibus*. Credo che non si possa continuare così. Questo crea poi dei nervosismi in Commissione che fanno togliere la parola dalla Presidenza a un senatore che stava intervenendo per una illustrazione; francamente per il nostro Gruppo è inaccettabile quanto accaduto oggi con il senatore Scarpinato. *(Applausi)*. intervengo per chiedere, a nome di tutto il Gruppo Partito Democratico, di far presente alla Presidenza intera che qui abbiamo bisogno davvero di un *time out* sulle modalità con cui si va avanti. Il senatore Balboni oggi ha aperto il vaso; della situazione, in ogni Commissione si toccano con mano le contraddizioni quotidiane di questo modo di fare, ma francamente non c'era mai successo, signor presidente Gasparri, di ritrovarci nella condizione di una decretazione d'urgenza *omnibus* (ci sono stati tanti che interviene con altri emendamenti del Governo su temi che nello stesso momento si stanno trattando con disegni di legge. È esattamente quello che richiamava prima il collega Scalfarotto e che è stato poi ribadito dal presidente Patuanelli. Siamo alla schizofrenia legislativa. Siamo ben oltre il monocameralismo alternato che di fatto ormai c'è ed è anche di pessimo livello.

vengono ratificate e spesso cancellano norme che si trovano in altri provvedimenti sempre proposti dalla maggioranza. Ormai c'è una competizione tra disegni di legge e decreti-legge. Una cosa simile francamente non la ricordo. presidente Gasparri, le chiediamo di informare il presidente La Russa e mi auguro che nella prossima Conferenza dei Capigruppo si possa affrontare seriamente questo tema partendo dall'intervento del senatore Balboni.

le sollecitazioni del presidente Balboni sono assolutamente pertinenti e quindi anche doveroso il dibattito che ne è seguito, è pur vero che si arriva a questa decretazione perché si sono affrontate esigenze esigenze di modifica normativa che molto spesso sono state trascurate in passato. Il decreto-legge oggi in discussione affronta sostanzialmente dieci specifiche problematiche, dieci specifiche criticità che, *a latere* di ogni retorica, costituiscono, comunque, mancanze che si sono consumate nelle precedenti legislature. Perché piaccia o non piaccia a qualcuno - considerando che gli italiani non si sono mai espressi chiaramente come in questa occasione a favore del centrodestra con il voto popolare - quelle forze politiche che avevano precedentemente governato non avevano inteso affrontarle. Infatti, questo decreto è stato terreno di discussioni, per lo più strumentali, dovute spesso a letture superficiali e semplicistiche dell'impianto normativo in questione, il cui fulcro, invece, sono norme fortemente volute da Fratelli d'Italia proprio per il contrasto alla criminalità organizzata e anche in ordine al rafforzamento delle norme di prevenzione. Il provvedimento si compone di tredici articoli. C'è l'introduzione di disposizioni in materia di processo penale e questo per una serie di finalità: consentire un efficace svolgimento del processo rispetto ad alcune tipologie delittuose e per rendere efficiente e sicura l'attività di intercettazione, garantendo i più alti *standard* di capacità investigativa rispetto a fattispecie di reato di particolare gravità; garantire un più celere svolgimento dei processi civili davanti al tribunale per i minorenni; dettare disposizioni sui corsi di formazione per il personale della magistratura; consolidare e rafforzare il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi in ragione della recente recrudescenza di episodi gravi e allarmanti; prevedere specifici interventi volti anche al recupero delle tossicodipendenze e di altre dipendenze patologiche; abolire gli obblighi a distanza di tanto tempo, - prima o poi qualcuno lo doveva fare - in materia di isolamento e autosorveglianza e modificare la disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica Covid; rivedere l'assetto organizzativo del Ministero della cultura e dettare disposizioni urgenti proprio per la cultura; dettare misure per garantire l'efficienza della pubblica amministrazione. Vedete, sono dieci specifiche finalità che nella loro obiettività costituiscono singoli momenti di particolare importanza nelle materie in cui esse incidono, così da palesarsi in un contesto di necessità e urgenza di intervento su temi fondamentali e di particolare importanza per l'Italia. Entrando nel merito delle disposizioni di legge, l'articolo 1 affronta il tema delle intercettazioni, attualmente contemplate per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia con il mezzo del telefono, prevedendo che le condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse si applichino anche ai delitti consumati o tentati di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di sequestro di persona a scopo di estorsione o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. Se chi lotta ogni giorno contro la criminalità organizzata lancia un grido di aiuto, ho la certezza che le norme che saremo chiamati ad approvare rispondono compiutamente a questo grido d'aiuto. Il Governo Meloni, dinanzi al grido d'aiuto dello Stato, risponderà sempre

dove la criminalità organizzata è riuscita a coniugare nel tempo una criminalità di natura primordiale con una criminalità che arriva a utilizzare la tecnologia più avanzata. Allora, se chi difende lo Stato ha l'esigenza di operare avendo a disposizione elevati e uniformi livelli di sicurezza e aggiornamento tecnologico,

dalle dichiarazioni del prossimo anno il settore delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche potrà contare sulla quota di 8 per mille statale direttamente assegnata dai cittadini. I dati ci dicono che c'è un'emergenza droga in Italia, che sembra essere stata catapultata nuovamente in una situazione simile a quella degli anni Novanta, con l'eroina che mieteva decine di migliaia di vittime, a cui si aggiungono l'uso sempre più diffuso di cocaina e droghe sintetiche (penso all'emergenza *crack* in molte delle nostre città)

Nel 2022 si è osservato un generale aumento dei consumi, che sono tornati a valori in linea o superiori rispetto addirittura a quelli prepandemici. Un'altra decisione importante presa dal Governo Meloni è quella di estendere la possibilità di destinare l'8 per mille al recupero delle tossicodipendenze e speriamo che questa opzione raccolga il favore di tutti coloro che non hanno mai voluto scegliere a chi destinare la propria quota. Lo dobbiamo a noi, ai nostri ragazzi e alle molte famiglie impossibilitate a sostenere i costi, spesso onerosi, legati ai percorsi di recupero di un familiare tossicodipendente, con problemi di alcol o ludopatico, consentendo loro di farlo. Vorrei, infine, soffermarmi su un punto del provvedimento che mi sta particolarmente a cuore: l'articolo 6, che apporta modifiche al reato di incendio boschivo. Il testo aumenta il minimo edittale della pena, sia nel caso si integri la fattispecie colposa che quella dolosa, prevedendo poi un'aggravante a effetto speciale nel caso in cui tale fattispecie sia commessa con abuso di poteri o violazione dei propri doveri inerenti la prevenzione e il contrasto degli incendi, o al fine di trarne profitto. Solo questa estate a Palermo, come a Catania e in molte altre città della Sicilia e del Sud Italia, ci sono stati centinaia, se non migliaia, di incendi. Un bilancio grave e una situazione particolarmente critica si registra soprattutto a Palermo, dove i danni degli incendi boschivi delle aree urbane si aggiungono a quelli della discarica cittadina di Bellolampo.

Un uomo di settantanove anni è stato fermato per aver appiccato un incendio ad Enna ed ha tentato di corrompere un carabiniere, offrendogli soldi per non proseguire l'indagine. Le procure di Foggia e Lecce hanno aperto fascicoli per incendio boschivo doloso per indagare sul rogo che ha distrutto 200 ettari nella baia di San Felice a Vieste.

In Sicilia, una delle Regioni italiane più colpite dai roghi estivi, la Regione, nel piano antincendio boschivo del 2020, parlava di un'industria del fuoco, cioè delle fiamme appiccate volontariamente per creare posti di lavoro nelle attività di avvistamento, di estinzione e nelle attività successive di ricostituzione. Anche gli incendi appiccati come protesta contro la mancata assunzione o come estrema forma di dissenso contro la minacciata chiusura di cantieri rientrano in questa logica, in cui il bosco assume ruolo di ostaggio. Tra le altre motivazioni che armano i piromani viene inclusa anche la volontà di eliminare i boschi per accaparrarsi terreni da coltivare o destinare al pascolo, in modo da intercettare i redditizi contributi comunitari o la volontà di trasformare aree rurali in aree edificabili. antimafia e della direzione nazionale antimafia hanno evidenziato come gli incendi siano legati spesso anche al ciclo dei rifiuti, su cui si allungano i tentacoli delle cosche. In particolare, capita che i rifiuti vengano stoccati in siti abusivi e poi smaltiti dandoli alle fiamme, con il rischio di generare roghi più estesi. Ma anche negli impianti di trattamento regolarmente autorizzati si verificano reiterate violazioni delle prescrizioni al fine di alleggerirsi del carico dei rifiuti incamerati. In Italia ogni anno, in media, secondo i dati del «Corriere della Sera», finiscono in manette tra piromani, cioè le persone con l'ossessione malata del fuoco e dei suoi effetti (la minoranza), e incendiari, cioè chi per colpa o per dolo appicca le fiamme da cui si propagano gli incendi boschivi. Noi siamo intervenuti - visto che qualcuno non lo ha fatto prima, perché alla fine sarebbe stato sufficiente scorrere le cronache giornalistiche per vedere che ogni anno questo Paese bruciava - e lo facciamo perché siamo favorevoli all'inasprimento delle pene per i piromani, sia per gli incendi dolosi che per quelli colposi. Gli incendi possono causare danni devastanti all'ambiente, alla flora, alla fauna e alla proprietà privata. Aumentare la pena minima da quattro a sei anni per gli incendi dolosi e da uno a due anni per quelli colposi è una misura adeguata a scoraggiare tali azioni irresponsabili e chi finora l'ha fatta franca, per proteggere il nostro patrimonio naturale e culturale. Inoltre, è importante garantire una giustizia equa e tempestiva per coloro che hanno subito danni a causa degli incendi, in modo da ridurre il rischio di impunità e incoraggiare il rispetto delle leggi a tutela dell'ambiente. Con l'occasione, esprimiamo ancora una volta la nostra profonda gratitudine ai Vigili del fuoco e alle Forze dell'ordine che si sono impegnati nei vari territori nelle attività di spegnimento e sostegno alla popolazione colpita dai roghi. Ancora una volta, il Governo Meloni è intervenuto e ci ha messo la faccia, segnando una vera inversione di rotta rispetto al passato. Presidente, vorrei richiamare l'attenzione sua e dell'Assemblea

Il provvedimento si compone di tredici articoli. Che cosa disciplina? Quali casi straordinari di necessità e urgenza intende affrontare? I primi due articoli si occupano di intercettazioni e intervengono su una materia estremamente complessa, che ha visto susseguirsi negli ultimi tempi diversi interventi legislativi. L'articolo 2-*bis* interviene invece in materia di contrasto alla criminalità informatica e in tema di cybersicurezza. L'articolo 3, invece, si occupa delle competenze che possono essere attribuite al giudice onorario da parte del tribunale dei minorenni. L'articolo 4 si occupa dei corsi di formazione per accedere agli incarichi semidirettivi e direttivi della magistratura. L'articolo 5-*bis* riguarda la dirigenza penitenziaria. L'articolo 6 interviene sulla disciplina dei reati a tutela del patrimonio boschivo. L'articolo 6-*bis*, già ricordato, introduce una nuova fattispecie di reato a tutela dell'orso bruno marsicano. L'articolo 6-*ter* interviene sulle responsabilità amministrative di coloro che sono preposti alla tutela dell'ambiente. L'articolo 7 si occupa di ridisciplinare parte della legge che regola la destinazione delle risorse raccolte

e che non siano state optate, cioè che i cittadini non abbiano espressamente indicato per quale tipo di destinazioni debbano essere impiegate, siano prioritariamente destinate al recupero della tossicodipendenza.

L'articolo 9 interviene sull'abolizione delle misure di isolamento e autosorveglianza e della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

nell'articolo 10 si proroga l'incremento del costo dei biglietti di ingresso nei luoghi e negli istituti di cultura. L'articolo 11 disciplina la possibilità di trattenere in servizio i dirigenti che hanno superato il limite di età, mentre l'articolo 11, comma 3-*bis*, si occupa di una particolare riserva nei concorsi degli enti locali. Non mi sono soffermato sulle specifiche dei vari commi, perché poi ogni articolo si occupa, nei diversi commi, di aspetti che non sempre sono collegati a ciò che è regolato nei commi successivi. la domanda che vorrei sottoporvi e che vorrei che tutti quanti ci ponessimo è: qual è la matrice razionalmente unitaria di questo decreto-legge? Che cosa accomuna la disciplina contenuta nelle diverse disposizioni che lo compongono? A me sembra poco o nulla; eppure, come sappiamo bene come sapete anche voi, la Corte costituzionale, in una giurisprudenza oramai consolidata, ha sottolineato come il decreto-legge, per essere conforme alla Costituzione, debba presentare un contenuto omogeneo: un decreto, una questione. La seconda domanda che vorrei che ci ponessimo è: i casi che vengono regolati sono straordinari e di necessità e urgenza? Ci sono i presupposti di cui all'articolo 77 per adottare questo decreto? Capisco che si voglia intervenire sulla destinazione prioritaria di una quota delle risorse reperite attraverso l'8 per mille per

per fare uscire le persone dalla tossicodipendenza? Questo è un caso straordinario che non era possibile prevedere, come una calamità naturale o un terremoto? *(Applausi)*. Ho fatto questo esempio, ma vale per tutte le disposizioni. È davvero difficile trovare un presupposto di necessità e urgenza straordinario, come pure la Costituzione prescrive. Vi è poi la procedura: la la legge di conversione è stata incardinata ieri alle ore 14 e alle 17,30 sono scaduti i termini per gli emendamenti. Questa mattina siamo in Aula dopo aver dedicato ben cinquantacinque minuti alla discussione, all'illustrazione, alla trattazione e alla votazione degli emendamenti. Persino il Presidente di Commissione, intervenuto in apertura dei lavori, ha sentito il dovere di denunciare

non sono un nostro privilegio, ma una funzione che la Costituzione ci obbliga ad esercitare. Rivendicare l'esercizio delle prerogative parlamentari significa adempiere a un dovere costituzionale. prima che sia troppo tardi e prima di ipotizzare stravaganti riforme costituzionali e improbabili elezioni dirette del Presidente del Consiglio, che non farebbero altro che peggiorare la torsione e la deriva che stiamo tutti sperimentando...

anomalo rispetto a quelli presentati anche da tanti Governi precedenti. Purtroppo - e lo dico con rammarico - ci troviamo di fronte a questo genere di provvedimenti urgenti senza poterli approfondire come il Parlamento dovrebbe, però è un'usanza ripetuta: i Governi

L'articolo 10 in particolare, di cui mi occupo, che riguarda il Ministero della cultura, ha infatti svariati commi e in quelli iniziali si parla soprattutto di una diversa organizzazione interna del Ministero, che ha una data (cioè va fatta entro il 31 dicembre 2023). L'organizzazione che si è data il Ministero della cultura è analoga a quella degli altri Ministeri e la segue, quindi abbandona l'organizzazione del segretario unico e prevede la suddivisione fino a quattro dipartimenti. Anche questa non è una cosa rivoluzionaria né nuova, perché quasi tutti i Ministeri sono organizzati in questo modo; erano rimasti in pochi a fare anche il Mistero della cultura ha fatto tale scelta di razionalizzare e cercare di fluidificare maggiormente la catena di comando per dare migliori risposte in termini di efficienza.

quasi dieci anni fa dal ministro Franceschini, intende invece compiere un passo verso una nuova fase della gestione dei luoghi della cultura e in particolare dei musei. Non si tratta solo dell'aumento da 44 a 60 istituti autonomi

Infatti, con le parole del ministro Sangiuliano, che mi preme ripetere, da oggi i grandi musei devono diventare piccole aziende: questa cosa farà storcere il naso a qualcuno, ma questi musei dovranno avere un modello gestionale che sia anche un po' imprenditoriale, il che non significa non garantire la salvaguardia storica del sito. Si ribadisce la procedura pubblica per selezionare i *manager* di alto livello, ma, come dicevo prima, a storici e professionisti di elevato livello culturale culturale si affianca chi ha esperienza nella gestione di enti, strutture e organismi pubblici e privati. Si apre quindi a un concetto più manageriale, che consenta alle organizzazioni complesse decisioni più rapide per migliorare la fruibilità, sempre nell'ottica di conservazione e di valorizzazione dei grandi siti culturali italiani, ovviamente sempre volte a perseguire scopi di natura pubblica, senza mai avere logiche di profitto. Il museo, quindi, è considerato non più esclusivamente un contenitore pregevole di beni culturali, ma un vero e proprio istituto culturale al servizio della società. Basti pensare che si parla di musei o parchi archeologici che potranno avere - sì - autonomia amministrativa (quindi la gestione del proprio patrimonio), ma che dovranno occuparsi non solo di conservazione, ma anche della parte espositiva, didattica, formativa. Si tratta di un sistema molto complesso di funzioni (basti pensare allo studio, alla didattica, alla ricerca, al *marketing*, al *fundraising*, ai servizi e ai rapporti con il pubblico, alle pubbliche relazioni, alle finanze e alla gestione di risorse umane, di strutture, di allestimenti e sicurezza), tra cui anche la valutazione, al passo con i tempi, degli investimenti tecnologici per la sicurezza la gestione delle autorizzazioni per l'utilizzo delle immagini dei beni che loro stessi custodiscono. Inoltre occorre ovviamente una dimestichezza con bandi e contratti per esternalizzare, laddove le professionalità presenti negli organigrammi dei musei non fossero all'altezza dei servizi concessi dagli istituti culturali degli altri Paesi. Tutto questo ovviamente senza perdere la vera *mission* del direttore del museo, ossia l'attuazione e lo sviluppo un progetto culturale e scientifico. Non a caso i direttori sono affiancati non solo da consigli d'amministrazione, ma anche da comitati scientifici, per mettere a terra una visione culturale e non solo manageriale. quindi dell'evoluzione di un ruolo dirigenziale molto composito, che deve conciliare la visione culturale con quella della pratica quotidiana, fatta di buona amministrazione, anzi di buona pubblica amministrazione.

al fine di contribuire alla ricostruzione del patrimonio culturale colpito dalle recenti alluvioni. Come sapete, la norma era scaduta il 15 settembre

con il Pantheon, qui vicino a noi, nei mesi di luglio e agosto abbiamo devoluto quasi 400.000 euro, in due mesi per un unico istituto statale, ma pensate che nel nostro Paese ce ne sono più di 4.000. Si comprende quindi l'importanza e l'urgenza di prolungare,

prima di entrare nel merito dei contenuti di questo ennesimo decreto-legge *omnibus*, di cui poi dirò cosa penso, desidero partire dalle parole del collega Scalfarotto e degli altri colleghi che mi hanno preceduto. Qui, colleghe e colleghi, dobbiamo decidere se ha ancora un senso la nostra funzione di parlamentari dentro quest'Aula. Le parole del presidente Balboni (e non è la prima volta) sono state molto chiare. chiare. Quali sono le prerogative di un senatore in quest'Aula? Sono quelle di poter vedere, leggere, studiare, preparare gli emendamenti ad un decreto-legge. Un decreto che, oltretutto, come ho detto, è l'ennesimo decreto *omnibus*

in maniera molto netta e molto chiara. Dunque mi domando, rivolgendomi soprattutto alla maggioranza, anche riprendendo le parole del collega Marcheschi, che mi ha preceduto: qual è, collega, la nostra funzione oggi? Perché può capitare, ed è capitato anche in passato, certamente, di avere dei decreti d'urgenza, dei decreti approvati con il voto di fiducia, ma non è mai successo di avere così poco tempo come quello che abbiamo avuto questa volta. Questo decreto è stato licenziato dalla Camera giovedì 28 settembre ed è arrivato in Senato ieri pomeriggio.

La premessa è d'obbligo: dobbiamo decidere cosa si vuole fare del lavoro dei parlamentari. Io credo che la dignità che sto rivendicando, e che altri colleghi stanno rivendicando in quest'Aula,

parlamentari e noi diventiamo quelli che devono soltanto ratificare un provvedimento. È evidente che non si può continuare così. Dobbiamo darci delle regole diverse. abbiamo già visto anche i precedenti decreti-legge: non solo decreti *omnibus*, cui ci ha abituato il Governo in quest'ultimo periodo, ma decreti che addirittura mettono insieme contenuti che non hanno nessuna nessuna possibilità di essere discussi contemporaneamente. Qui si va dall'orso marsicano a san Francesco e a norme penali, quindi andiamo a legiferare su un tema delicatissimo relativo alla giustizia senza avere tempo neanche di leggere il provvedimento. Vorrei chiedere a quest'Aula chi ha avuto la possibilità di studiare questo provvedimento. Io, da senatrice,

Presidente, rivolgo anche a lei questo appello, perché deve essere chiara la funzione, che noi dobbiamo rivendicare, con le nostre prerogative costituzionali di parlamentari *(Applausi)* e la difesa della democrazia parlamentare, almeno fino a quando ci sarà il Parlamento. Parlamento. Colleghi, entro nel merito di questo provvedimento, ovviamente facendo finta di aver avuto il tempo necessario per approfondirlo.

o di ostilità nei confronti del Governo. Come sapete, soprattutto in materia di giustizia e di intercettazioni, abbiamo sempre voluto discutere nel merito. Io ringrazio sempre il collega Scalfarotto per l'ottimo lavoro che sta portando avanti nella Commissione competente,

Sono molto preoccupata, perché stiamo andando a legiferare appunto su materie che riguardano il personale della magistratura e della pubblica amministrazione, salute, la cultura, il recupero della tossicodipendenza, il contrasto agli incendi boschivi e disposizioni urgenti in materia penale. Io non credo che questo sia un modo di lavorare correttamente. Poi, certo, all'interno del dei passi assolutamente importanti, in modo particolare il contrasto alla criminalità e il rafforzamento della difesa dei soggetti pubblici e privati rispetto a tutto il tema legato alla criminalità informatica alla cybersicurezza. Però ci sono degli emendamenti che non hanno potuto essere visionati dalle Commissioni congiunte, su cui avremmo potuto dire la nostra e avere anche magari un voto unanime da parte delle Commissioni. Invece siamo in Aula senza relatore e senza aver discusso minimamente nessun tipo di emendamento. È chiaro quindi che il nostro è un giudizio profondamente negativo: nel merito, nell'atteggiamento, nel metodo di questo Governo e anche perché siamo qui a difendere prima di tutto la dignità del lavoro parlamentare di maggioranza e di minoranza. Concludo dicendo che poi il collega Scalfarotto, in dichiarazione di voto, di voto, dirà ancora di più nel merito quello che è accaduto in queste poche ore che abbiamo avuto a disposizione. Rimane agli atti che che da parte nostra ci sarà un voto contrario su questo decreto, prima di tutto per il metodo che ancora una volta è stato adottato da questo Governo.

il decreto-legge che andiamo ad esaminare oggi e a convertire in legge è stato approvato, come ben sappiamo, il 7 agosto dal Consiglio dei ministri. Poi è stato presentato alla Camera dei deputati, dove è stato esaminato a lungo.

hanno valutato e approfondito i diversi temi che il decreto tratta. Sulla parte che riguarda le tematiche della giustizia interverrà dopo per il nostro Gruppo, per competenza, il senatore Zanettin. Voglio solo dire, da siciliana, che sulla lotta alla mafia Forza Italia ha una storia trentennale in Parlamento, di cui parlano gli atti e le norme adottate e di cui vado fiera, dalla confisca allargata dei beni ai mafiosi al carcere duro per i capimafia, all'aumento dei poteri del procuratore nazionale antimafia (solo per citare alcune misure normative che dobbiamo al presidente Berlusconi) e all'importante attività dei Gruppi parlamentari di Forza Italia, attraverso l'adozione di strumenti con i quali sono stati arrestati migliaia di mafiosi, sequestrati miliardi di euro di beni e rese inefficaci le loro azioni criminali. Dico questo, perché si è tentato di strumentalizzare la parte del decreto al nostro esame che riguarda le intercettazioni ambientali, bollandola come un favore ai mafiosi. Bene, nessun favore ai mafiosi; anzi, le fattispecie in cui viene applicata la disciplina delle intercettazioni vengono ampliate a reati come il traffico illecito di rifiuti, che oggi è proprio uno dei nuovi redditizi *business* della criminalità mafiosa. A tal proposito, voglio ricordare che alla Camera è stato persino aggiunto un articolo al decreto che inasprisce il trattamento sanzionatorio in materia di delitti contro l'ambiente. L'intervento normativo previsto dal decreto sulle intercettazioni a strascico ripristina quelle garanzie individuali che anni di divulgazione di conversazioni riguardanti persone non coinvolte in fatti criminali hanno calpestato. Le nuove norme bloccano la gogna mediatica, ma non fermano le indagini, soprattutto nei confronti dei criminali. Non si potranno trascrivere quelle intercettazioni che riguardano fattispecie diverse da quelle dei reati per cui invece si indaga. Chiaramente sono esclusi i reati gravi, per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, così come sono esclusi i reati di mafia e di terrorismo. Questa è la mia sintesi, quello che capisco io e che capiscono le persone di buon senso. Sulla questione, come ho detto poc'anzi, il collega Zanettin sarà certamente più preciso soprattutto sui termini tecnico-giuridici. Altro tema sul quale intervengo è il reato di incendio boschivo. Il provvedimento, come già ricordato, è stato adottato ad inizio agosto, proprio mentre la Sicilia veniva devastata da una serie di incendi. I danni, come sappiamo tutti, sono stati enormi non solo per l'ambiente e per il territorio; hanno subito danni infatti

Sono state interessate anche molte strutture civili. Il decreto-legge contiene una norma che aumenta la pena minima edittale prevista dal codice penale sia nelle ipotesi di delitto doloso che in quelle di delitto colposo. Viene introdotta l'aggravante nel caso in cui il reato sia commesso con abuso di potere o violazione dei propri doveri di prevenzione. Spesso infatti è chi deve vigilare che appicca i fuochi o fa finta di non vedere. Si introduce quindi un nuovo quadro giuridico che farà riflettere chi vuole speculare o guadagnare attraverso gli incendi boschivi. Vorrei concludere ricordando che il decreto-legge contiene molte altre misure puntuali; dalla destinazione dell'8 per mille alle disposizioni sulle PA, ben evidenziate nel corso del dibattito svoltosi alla Camera dei deputati. Ancora una volta siamo di fronte a un decreto-legge che va nella direzione di attuare un programma di centrodestra che si svilupperà nel corso dell'intera legislatura, mettendo quindi mano con costanza a tutte quelle norme che rallentano lo sviluppo di questo Paese. *(Applausi)*. Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, prendendo spunto dalle parole del maestro Battisti, dico «Ancora tu». L'Assemblea è chiamata a convertire l'ennesimo decreto-legge; ormai ne abbiamo perso il conto.

Solo analizzando il titolo del decreto-legge perderei la metà del tempo relativo al mio intervento. Credetemi sulla parola: non è né omogeneo né rispettoso dei citati requisiti. Il mio intervento verterà sulle questioni di stretta attinenza alla Commissione giustizia. Articolo 1: il decreto-legge nasce dall'esigenza di creare una norma di interpretazione autentica volta al superamento di una sentenza di una sezione semplice della Cassazione che escludeva l'applicazione del meno severo regime di autorizzazione alle intercettazioni per i diritti di criminalità organizzata per i reati monosoggettivi ancorché realizzati con l'aggravante di mafiosità,

Se l'intento era quello di creare una norma di interpretazione autentica, avete disposto una norma che a prima lettura sembrerebbe invece una norma procedimentale. Bene, sappiamo noi, ma sono certa anche voi, che le norme di interpretazione autentica non necessitano di norme transitorie, ma sono di per sé applicabili retroattivamente. Perché allora non approvare il nostro emendamento, presentato anche in sede di esame alla Camera, che prevede una norma di interpretazione autentica e, quindi, applicabile anche ai procedimenti in corso? Invece di semplificare la questione con questa norma, l'avete complicata.

Aula, tramite il Presidente del Senato - abbiamo appena concluso, fin dalla modifica richiesta dal senatore Zanettin, una proficua indagine conoscitiva sulle intercettazioni. Perché secondo lei la maggioranza ha voluto mortificare l'indagine conoscitiva facendo approvare emendamenti che annacquano tutto il lavoro svolto dalla Commissione e anche - devo dire - il lavoro svolto dal presidente Bongiorno? Ci sono vari punti sul tema che vorrei toccare. Il primo è

Cosa si intenda per autonoma valutazione non è dato sapersi: l'autonomia va intesa quale differente e/o ulteriore rispetto a quella del pubblico ministero? Uguale, ma con parole diverse? Siamo veramente al teatro dell'assurdo. Il secondo punto è la mancata trascrizione, neanche sommaria, delle intercettazioni considerate *prima facie* come irrilevanti. Tutti in quest'Aula sappiamo che i brogliacci li fa la tutti noi conosciamo la mole di lavoro che c'è per portare all'attenzione del pubblico ministero l'ingente materiale intercettato, il che vuol dire che l'attività di selezione del materiale è disposta da molteplici operatori, i quali, non potendo avere contezza dell'intero materiale, selezionano ciò che a prima vista potrebbe reputarsi necessario. Non essendo riportati nei verbali né nelle annotazioni, sarà impossibile per l'avvocato riuscire a reperire elementi a favore dell'indagato, il quale vedrà compromesso il proprio diritto di difesa. C'è un ulteriore tema sul quale richiamo ancora l'attenzione della presidente Bongiorno. In Commissione abbiamo appurato da un lato che i costi delle intercettazioni sono in costante diminuzione rispetto anche al passato prossimo e dall'altro abbiamo constatato l'ingente ritorno economico delle stesse in ragione dei provvedimenti ablatori disposti grazie al loro utilizzo. Il saldo, in questo caso, è attivo. Grazie alle intercettazioni, lo Stato acquisisce ricchezza, non la disperde. che però è il più importante, è quello della modifica relativa alle cosiddette intercettazioni a strascico. Letta in questo modo, potrebbe sembrare anche una modifica innocua e forse anche sentita dagli interpreti, ma nulla è più sbagliato. Con questa norma si intende escludere la possibilità di utilizzare le intercettazioni disposte per un determinato procedimento in un altro, fatta eccezione per i reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Prima dell'intervento del Governo, oltre a quanto già detto, i risultati delle intercettazioni potevano essere utilizzati in altri procedimenti se aventi ad oggetto delitti rientranti tra quelli per i quali le intercettazioni potevano essere disposte. Cosa cambia? Che prima dell'intervento del Governo era possibile utilizzare le intercettazioni in altri procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione, mentre adesso no. Chiaro? Sempre in tema di giustizia, occorre segnalare due disposizioni che critichiamo per la medesima *ratio*: le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni e le disposizioni urgenti in materia di contrasto alla criminalità organizzata e di cybersicurezza, la prima inserita nel decreto, la seconda invece con un emendamento governativo alla Camera. Ma ci rendiamo conto? Temi così importanti inseriti in un decreto nottetempo, con tempi di esame così contingentati?

Intervenite su questioni che attengono alla sicurezza nazionale in maniera assolutamente scellerata. Su tali temi serve concertazione, serve uno studio approfondito, serve tempo. Sul tema degli incendi, perché dare parere contrario alla Camera - questo me lo dovete proprio spiegare - su un emendamento che dispone l'interdizione perpetua dai pubblici uffici nei confronti di coloro che si macchiano per tali ignobili condotte?

Anche questa volta il Parlamento sarà mortificato dall'ennesima fiducia. Ricordiamo con stupore e rimpianto lo sgolarsi dell'onorevole Meloni che tacciava la maggioranza di governare con decreti-legge; lei, espressione del Governo che ha utilizzato di più lo strumento della decretazione d'urgenza rispetto a tutti gli altri Esecutivi della storia repubblicana, figuriamoci se avesse dovuto gestire l'emergenza Covid, non voglio nemmeno pensare a quanti ne avrebbe prodotti. Ci troviamo di fronte all'ennesimo provvedimento che mette in luce le due visioni della giustizia all'interno della maggioranza: garantisti e giustizialisti. Il risultato è l'ennesima lenzuolata di norme valevoli dalla sera alla mattina, che saranno impugnate dalla Consulta mortificate sicuramente nel futuro prossimo. Vorrei formulare un ultimo invito in riferimento alla gestione dei lavori di Commissione, dopo quello che è successo oggi. Io capisco le questioni politiche e i punti di vista,

ad un senatore di illustrare un proprio emendamento, in quanto non veloce nel ricercare lo stesso nel fascicolo *(Applausi)*; fascicolo che, ripeto, è giunto solo poco prima che iniziasse la seduta della Commissione stessa. Lo trovo assurdo, signor Presidente.

da questo Governo, che dal suo insediamento si è gloriato di dire che è un Governo politico e che la Presidente del Consiglio è stata lei stessa parlamentare per anni e quindi ha sommo rispetto del ruolo del Parlamento.

autoritaria e arrogante, con la mancanza di rispetto della dignità dei colleghi e delle colleghe presenti, al punto da togliere loro la parola nel pochissimo tempo che avevano a disposizione. Invito

Grazie

redazionale di un testo che (spiegherò tra poco nel dettaglio per quali ragioni) ha dovuto occuparsi di materie apparentemente non troppo collegate tra loro, ma che, in uno spirito che questa maggioranza e questo Governo avevano annunciato sin dall'inizio, va nella direzione di diminuire il grado di influenza della burocrazia di fornire norme aggiornate al presente e, non ultima, una migliore organizzazione delle figure apicali che si occupano di settori strategici per il nostro Paese. nostro Paese. Si va dalla materia penitenziaria fino a toccare anche quella del Ministero dei beni culturali, con un riordino delle aree funzionali; si tocca addirittura anche quella dei dirigenti generali, delle direzioni, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti.

i rincari dei materiali e dell'energia e stiamo continuando a destinare risorse all'emergenza energetica. Quotidianamente,

utilizzare in maniera più intelligente le risorse di cui abbiamo gran bisogno. Tra queste, ad esempio, la necessità di poter utilizzare, per incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, personale che magari non è più al lavoro. di evitare di doverlo attingere da strutture amministrative, distogliendo energie e competenze da quelle strutture che in questo momento sono destinate a concretizzare le progettualità del PNRR, su cui abbiamo delle difficoltà temporali. La grande capacità ingegneristica è magari minata dalla difficoltà di reperire anche le competenze: abbiamo visto quanto sia complesso fornire alle imprese non tanto e non solo gli operai, ma anche figure tecniche specializzate che non si trovano con la bacchetta magica, e spesso e volentieri sono reperibili all'estero. È per questo che il Governo ha intelligentemente ampliato la possibilità di far ricorso a quella immigrazione legale di cui abbiamo bisogno, e non a quella proveniente in maniera del tutto irregolare da situazioni

focalizzare l'attenzione su alcune tra le norme che questo decreto-legge contiene. Ad esempio, vorrei citare l'attenzione alla repressione di condotte irresponsabili e dolose e dolose e l'incremento delle pene per i reati afferenti agli incendi. Abbiamo patito tutti sui nostri territori quanto possa

quelli siciliani e sardi dalle difficoltà conseguenti a un incendio avvenuto in piena stagione turistica. Vorrei citare anche i casi minori, come l'isola d'Elba. Pochi giorni fa, si è avuto uno dei primi casi, in provincia di Pisa, in cui si applicheranno queste norme di maggior rigore anche nei confronti di condotte colpose per aver cagionato un incendio, magari per disattenzione; ebbene, tali condotte un po' più alta. Speriamo di poter sensibilizzare in questo modo anche i cittadini a rispettare quell'ambiente che molto faticosamente siamo riusciti ad inserire anche tra i valori costituzionali di questo Paese. L'inasprimento del trattamento sanzionatorio va di pari passo con una altrettanto intelligente allocazione di risorse per rimediare agli effetti della terribile pandemia

la quota Irpef di competenza dello Stato qualora non ci siano state delle scelte espresse da parte del contribuente sulla destinazione di quelle somme. Che cosa si fa? Si destinano prioritariamente per la lotta alle tossicodipendenze e alle altre forme di dipendenze psicologiche. Sappiamo

qualcosa in più.

e sociale; dall'altra parte, garantire che alcuni degli strumenti utili all'intercettazione, come il captatore, possano venire utilizzati - lo deciderà il Governo attraverso decretazioni successive

di tali strumenti, citai il caso della captazione di una confessione religiosa, uno dei momenti sacrali nell'ambito della fede cristiano-cattolica. Evidentemente il captatore può entrare non solo nelle nostre abitazioni, ma anche in momenti di vita privata. Quindi, saranno previste delle garanzie - vado a concludere anche nei confronti di quei contenuti che sono del tutto irrilevanti ai fini dell'indagine per poterli espungere in maniera definitiva e certificata dal contenuto divulgabile per le successive fasi processuali, a garanzia della riservatezza e dell'integrità persone. Mi sento di anticipare quindi - poi sul resto, in sede di dichiarazione di voto, la collega Stefani potrà approfondire molto meglio del sottoscritto gli aspetti tecnici relativi all'utilizzo dell'intercettazione

Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi,

che sia tornata la politica vuol dire che c'è un Esecutivo che tutto determina e, prima ancora dell'opposizione,

con la questione delle garanzie in senso ampio che vengono spesso evocate, mi chiedo se la dittatura dell'Esecutivo e il suo ruolo preminente stiano in una cultura delle delle garanzie e nel rapporto con gli altri poteri dello Stato, ma tant'è. E sempre per parlare delle garanzie, uno dei pilastri e dei presupposti delle garanzie è la certezza del diritto. questo decreto-legge, che è iniziato su una questione interpretativa - per così dire - dopo una sentenza della Corte di cassazione che contraddiceva un orientamento delle sezioni unite, siamo partiti a discutere di Cassazione e siamo finiti sull'orso marsicano;

perché c'era la necessità di intervenire con urgenza dopo le esternazioni sul concorso esterno in reato mafioso del nostro ministro Nordio, e forse nella fretta si è persa di vista la coerenza normativa.

Se fosse una norma interpretativa, sarebbe ovvio che valeva in allora; adesso non si saprà e c'è una grande incertezza sul fatto che possa disciplinare anche le intercettazioni già fatte prima (e in questo caso verranno sollevate questioni di legittimità) o addirittura

oltre che essere un grande pasticcio, questo va chiaramente a incidere sulla certezza del diritto e guardate che di nuovo sta fuori dalla cultura delle garanzie.

su questioni che sono già state affrontate da importanti riforme; anziché pensare eventualmente di migliorarle, si fa come se non esistessero - importa di più fare qualcosa di molto ideologico

in quell'indagine conoscitiva, un punto su cui noi eravamo d'accordo riguardava l'archivio segreto in cui devono finire tutte le intercettazioni che non sono pubblicabili, ma sono fruibili dalla difesa per

Scusate: prendersi carico delle tossicodipendenze vuol dire che su fondi già destinati ad altre questioni di carattere sociale non si stanzia un euro in più, ma semplicemente si prevede

di rinvii e di aggiustamenti. Dite che non siete d'accordo, che non vi piace il contenuto fondamentale, che non vi piacciono le linee programmatiche di questi fondi, che sono coesione sociale, parità,

che ovviamente di colpo cesseranno solo per questo fatto. Vorrei concludere citando alcune parole del ministro Nordio sulla questione dell'aumento delle pene. Ma non vi citerò parole precedenti all'incarico del ministro Nordio. Vi cito un'intervista del 16 settembre 2023 a "Il Foglio", laddove, interpellato sull'aumento delle pene, dice: «Se si guardano gli aumenti delle pene sotto il profilo dell'efficacia preventiva del reato, confermo quello che ho detto: è illusorio pensare che un aggravamento delle pene funga da deterrente.

della sua attenzione verso la gravità di certi reati». E questo segnale lo Stato lo dà (e cito sempre l'intervista) «senza farsi l'illusione che la pena costituisca un deterrente. (...) Sotto questo profilo, l'aumento della pena ubbidisce al principio che nessuno cita mai: l'allarme sociale». E abbiamo liquidato così secoli di cultura liberale, di cui si affermano paladini questo Ministro e questa maggioranza, e siamo in un grandissimo e bellissimo populismo giudiziario.

come al solito si sfrutta un provvedimento in discussione per parlare di tutto e di più.

aggiungendo che non sono d'urgenza. Io vi faccio un esempio banale: un buco per strada nell'asfalto è manutenzione ordinaria. Cento buchi, causati dal non aver fatto interventi su quel buco, diventano manutenzione straordinaria. Se questo Governo e questa maggioranza, ad ogni lato del panorama verso cui si girano, trovano buchi normativi è per inefficienza oppure per non intervento di chi c'è stato prima. Allora siamo costretti, il Governo è costretto, a intervenire d'urgenza, laddove noi ci guardiamo e c'è bisogno di un provvedimento oppure quel provvedimento non c'è o è obsoleto oppure non è più al passo coi tempi. Ecco perché poi sorge la necessità, che io comprendo anche come critica, di partire con un provvedimento e di sommare poi in esso altre materie: tutte accomunate, però, dall'urgenza e questo è vero.

luogo, nessuno ci aveva mai pensato prima e quindi quei fondi chissà dove sarebbero andati. Noi, invece, diamo loro una finalità precisa. In secondo luogo, i soldi che c'erano, che i Governi precedenti avevano stanziato, non erano sufficienti, perché altrimenti non avremmo avuto bisogno di cercarne altri.

è la punta dell'*iceberg* di una periferia; quanto avviene nei boschetti attorno alle grandi città, a partire da Milano, ma anche a Roma, è sotto gli occhi di tutti da anni e nessuno è intervenuto su questo. Se serve la repressione, se serve punire chi spaccia, anche il piccolo spacciatore,

fumando o inalando la cocaina, ma si è tornati alle siringhe, che sono la cosa più pericolosa, anche dal punto di vista sanitario, lasciando da parte, ma non dimenticando, gli altri danni che le droghe Come ha detto l'altro giorno don Patriciello, audito dalle due Commissioni riunite, è necessario formare, educare, spiegare, ma è anche necessario reprimere. allora, all'altro argomento che ci avete contestato in Commissione e questa mattina in Aula. Voi dite che aumentare le pene risponde solo all'esigenza di dimostrarci forti con l'opinione pubblica? No: non serve solo a quello,

Bene, ma c'è un fine della pena, cui nessuno pensa mai e di cui nessuno parla mai, che è il fine speciale preventivo.

in uno dei due casi: per evitare che uno continui a fare i reati o per prevenire chi, pensando a quanto potrebbe pagare come pena, non lo fa più.

corrette e che su di esse non possiamo non essere concordi, anche laddove - e non lo ha citato nessuno - si inizia a dare un minimo di di attenzione ai *trojan*, spiegando come possono essere utilizzati. Penso che sia molto utile quello che è stato scritto nell'articolo 1. Inoltre, a riprova del fatto che non siamo meri esecutori di ordini del Governo

Pensiamo anche che la Camera abbia fatto un buon lavoro nel modificare il decreto. I tempi qua sono stati quello che sono stati; lo hanno già ribadito tutti e mi accomuno a quanto è stato detto. Ma non accettiamo l'accusa di essere meri notai di quello che fa il Governo. Non è così. Tornando alle intercettazioni, penso sia un grande passo in avanti il fatto che ci sia un archivio nazionale delle intercettazioni,

all'articolo 1, è un po' smontato quello che si dice, cioè che questa maggioranza sia contro le intercettazioni, perché - come vedete - ne abbiamo ampliato l'uso.

corrette. Il nostro intervento di oggi, che concludo per conto del mio partito, in attesa delle dichiarazioni di voto, non può che far salire, sopra il livello delle acque torbide che sotto si volevano dimostrare, quelle acque limpide che fanno luce su un decreto utile, compreso quello dell'orso, che tanti hanno deriso.

generale. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà. Signor Presidente, colleghi senatori, a nome del Governo e autorizzato dal Consiglio dei ministri pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi,

È una sorpresa e ve ne private. Presidente Zaffini, non si aggiunga. Cerchiamo di andare avanti e facciamo concludere in silenzio il ministro Ciriani. in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero

della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 105, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati. È convocata la Conferenza

una nuova finestra"). La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione del dibattito sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione del decreto-legge in materia di incendi boschivi, tossicodipendenze, salute e cultura, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, alle quali seguirà la chiama. La Conferenza dei Capigruppo ha altresì approvato il calendario dei lavori fino al 26 ottobre. Restano confermati, per la seduta di domani, il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*, con la presenza dei Ministri della difesa, dell'agricoltura e del lavoro. Il calendario della prossima settimana prevede la discussione dei disegni di legge istitutivi della Commissione parlamentare di inchiesta sull'emergenza SARS-CoV-2 e, dalla sede redigente, della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Orlandi e Gregori. Gli emendamenti al disegno di legge per l'istituzione della Commissione Covid dovranno essere presentati entro le ore 12 di venerdì 6 ottobre. Mercoledì 11 ottobre si discuterà l'autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Corrado Clini, in qualità di Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare *pro tempore*. Il risultato della votazione non verrà proclamato immediatamente poiché i senatori che non hanno partecipato alla votazione elettronica potranno dichiarare il proprio voto palese ai senatori Segretari fino alla chiusura delle operazioni di voto, prevista dopo il voto sulla NADEF. Sempre mercoledì 11 si discuteranno congiuntamente la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023 e l'annessa Relazione al Parlamento sullo scostamento dagli obiettivi programmatici di indebitamento. Per quest'ultima è necessario il voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Le proposte di risoluzione alla NADEF e alla Relazione annessa dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale. Gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 dovranno essere presentati entro mezz'ora dall'espressione del parere. Le votazioni sui documenti non avranno luogo prima delle ore 17. La settimana dal 16 al 20 ottobre sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle Commissioni. L'Assemblea si riunirà martedì 17 e, se necessario, mercoledì 18 ottobre, fino alle ore 13, per la discussione del decreto-legge su qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. Mercoledì 25 ottobre, alle ore 10, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre 2023. Nella stessa settimana si discuteranno le proposte di questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, sul decreto-legge per il contrasto del disagio giovanile. Seguirà la trattazione nel merito del provvedimento. Il calendario potrà essere integrato con il rendiconto 2022 e il bilancio interno 2023 del Senato e con la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato per resistere in un conflitto di attribuzione. Giovedì 12 e 26 ottobre avranno luogo il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*.

oggi è un giorno molto triste per il nostro Paese, in particolare per Mestre e per Venezia. Ieri sera, come ha ricordato questa mattina il Presidente, un viaggio che aveva condotto persone di diversa nazionalità a vivere momenti di gioia per visitare una tra le più belle città del mondo si è trasformato in una tragedia. È difficile trovare parole adeguate di fronte a ventuno morti, tra i quali bambini e adolescenti, e quindici feriti, alcuni molto gravi. Vogliamo esprimere qui il nostro cordoglio per le vittime, la vicinanza alle loro famiglie e l'augurio di pronta guarigione ai feriti e ringraziare al tempo stesso tutta la macchina dei soccorsi, a partire dai cittadini che per primi hanno segnalato l'incidente, per l'impegno profuso in queste ore non facili. Tutto il Veneto, con il personale sanitario, i Vigili del fuoco, le Forze dell'ordine, la Protezione civile, ha risposto con quella generosità e quella solidarietà che sono proprie dei veneti. È giusto che queste siano, in nome delle vittime, le ore del dolore e del silenzio. Arriverà il tempo per accertare la dinamica dei fatti, per capire cos'è realmente accaduto in quegli attimi drammatici. Nulla purtroppo ridarà la vita a chi l'ha perduta, ma la ricerca della verità è doverosa per rispettare la loro memoria e il dolore delle loro famiglie. Già oggi leggiamo ricostruzioni: è comprensibile che questo possa far parte del dovere di cronaca, è però opportuno attendere che le autorità chiamate a farlo, a partire dalla magistratura, possano procedere con mezzi e tempi adeguati in un contesto che consenta loro di operare al meglio. Tutte le istituzioni competenti saranno chiamate a svolgere la propria parte in questa ricerca della verità. Anche in questa sede, dal punto di vista parlamentare, ci attiveremo perché ciò possa avvenire. Mestre, Venezia, il Veneto e il Paese tutto oggi piangono le vittime. Ai loro familiari vada il nostro più sincero e profondo cordoglio.

voglio intervenire in questa sede per esprimere il cordoglio nostro e credo di tutto il Paese per questa immane tragedia che abbiamo appreso ieri sera

Non è questo il momento - com'è già stato detto prima di me - dell'accertamento delle responsabilità, ma credo che doverosamente chi è preposto a farlo svolgerà degli accertamenti per capire una dinamica che ad oggi appare inspiegabile rispetto a quanto a quanto accaduto, soprattutto per il suo esito disastroso in termini di perdita di vite umane e di feriti. Quindi, esprimo la solidarietà mia personale, della mia capogruppo, Licia Ronzulli, e di tutto il Gruppo Forza Italia alla città di Venezia, alla Regione Veneto,

ai messaggi di cordoglio espressi poco fa dai colleghi che mi hanno preceduto, nonché di vicinanza alle vittime del terribile incidente. È una tragedia che ci sconvolge e che purtroppo abbraccia

ci uniamo al cordoglio per le vittime ed esprimiamo vicinanza alle famiglie delle persone che stanno lottando per la sopravvivenza. Ringraziamo tutta la macchina dei soccorsi che si è attivata immediatamente, dai Vigili del fuoco alla Protezione civile, alle Forze dell'ordine al personale sanitario, che in queste ore sta lavorando per rendere meno tragica questa giornata. Nelle prossime ore

Per ora conosciamo solo un nome, quello di Alberto Rizzotto, il conducente: alla sua famiglia vanno la nostra vicinanza e il nostro cordoglio. È difficile trovare le parole, oggi: è anche il momento in cui tutti dobbiamo stare in silenzio, in attesa che le prossime ore rendano più chiara la dinamica. anche l'Amministrazione comunale e la Regione Veneto, perché so che si sta attivando anche per dare un supporto psicologico alle famiglie delle vittime che arriveranno da ogni parte d'Europa.

Signor Presidente, mi unisco al cordoglio nei confronti delle vittime e dei vicini veneti, perché, purtroppo, questa tragedia è appunto accaduta in Veneto. Voglio esprimere tutta la mia solidarietà alle Forze dell'ordine, ai militari, ai Vigili del fuoco, alle forze di soccorso, perché in queste ore stanno lavorando alacremente. Dal primo istante sono intervenuti

Voglio solidarizzare in particolar modo con la città di Venezia, col sindaco Brugnaro, che dal primo istante si è recato sul posto. Ha parlato, appunto, di una immane tragedia e ha indetto ovviamente il lutto cittadino. Anche in questo, le istituzioni si sono fatte trovare pronte, insieme al Presidente della Regione e a tutti gli operatori del soccorso. Spiace che questa tragedia sia avvenuta sul nostro territorio. Spero soltanto che non ci sia la corsa a capire di chi sono le colpe. È un tragico incidente stradale. Purtroppo dobbiamo pensare, in questo momento, soltanto alle vittime e pregare per loro.

nel corso degli anni non mi ha dato la percezione di essere un luogo sul quale si potesse poi raccontare una tragedia come quella che abbiamo vissuto, come comunità

la solidarietà ed una forte vicinanza nei confronti dei familiari e dei feriti che stanno cercando di uscire dalle terapie intensive e dalle sale degli ospedali. Chiaramente il ringraziamento, in questo momento, va a tutti coloro i quali sono intervenuti prontamente, ai cittadini che hanno segnalato quanto stava accadendo, ai Vigili del fuoco, che ieri sera hanno operato in condizioni estremamente difficili e sono e sono riusciti a salvare molte vite umane che, senza il pronto intervento da parte dei Vigili del fuoco e degli uomini della Protezione civile, probabilmente oggi sarebbero da annoverare nell'elenco drammatico Poi, oltre alle Forze dell'ordine, ringraziamo tutto il personale socio sanitario, che da ieri, mettendo in moto una macchina incredibile dal punto di vista organizzativo, ha garantito il ricovero immediato in tantissimi ospedali della Regione Veneto di tutte le persone coinvolte dall'incidente. Ovviamente la vicinanza del Gruppo Fratelli d'Italia va a tutti i familiari delle vittime e anche ai popoli delle Nazioni ai quali appartengono le vittime ed i feriti. Tra di loro c'erano, infatti, molti ucraini, c'erano spagnoli, francesi, tedeschi, croati, austriaci. Insomma, c'era un pezzo d'Europa all'interno di quel pullman. Verrà il momento e, anzi, prossimi giorni, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi ci saranno tutti gli accertamenti del caso, per capire quali sono state le ragioni che hanno portato a questa tragedia. In questo momento, quello che mi sento di dire è che ci stringiamo attorno al dolore dei familiari delle vittime, dei loro amici e anche dei loro connazionali e che ovviamente siamo vicini alla famiglia di Alberto Rizzotto, il nostro connazionale che ha perso la vita in occasione dell'incidente. Grazie a tutti. La Presidenza si associa al cordoglio e alla vicinanza espressa da tutti voi alle vittime. Già stamattina abbiamo ricordato le vittime nel minuto di silenzio che abbiamo osservato. Ringraziamo davvero tutti i soccorritori e le Forze dell'ordine.

Presidente, il decreto-legge n. 105 del 2023 reca disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute, di cultura e ancora in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. Chiaramente ci troviamo di fronte all'ennesimo decreto *omnibus*; è già il titolo che rende impossibile camuffarne la sua piena eterogeneità. Questa è quindi l'ennesima volta in cui il Parlamento è stato declassato da legislatore a organo di ratifica dei decreti dell'Esecutivo, sui quali, per di più, spesso e volentieri viene posta la questione di fiducia, per accelerarne l'approvazione e risolvere qualche problemino in maggioranza, incuranti del fatto che, così facendo, si svilisce completamente il ruolo del Parlamento. Se alcune delle questioni affrontate dal provvedimento possono considerarsi condivisibili (penso ad esempio all'articolo 1), nei lavori in Commissione alla Camera non c'è stata la possibilità di convincervi della pericolosità della formulazione del combinato disposto tra il primo e il secondo comma. Il dramma è quindi che la stesura ne ha annullato ogni effetto positivo e, come evidenziato da numerosi auditi alla Camera, il rischio è che questa norma, nata, nelle dichiarazioni di Governo, per risolvere una questione interpretativa, si riveli poi incostituzionale, aggiungendo quindi dubbi interpretativi e contenziosi e complicando quindi ulteriormente la situazione. Respinti dalla maggioranza tutti i tentativi di migliorarne il testo in fase emendativa, sono state approvate disposizioni che puntano chiaramente a indebolire la lotta contro la corruzione. Ci sembra infatti evidente che i provvedimenti che questo Governo ha in mente in tema di giustizia (le limitazioni poste all'uso delle intercettazioni e le modifiche alla disciplina sui collaboratori di giustizia da una parte, l'abolizione del reato di abuso d'ufficio dall'altra) siano tutti elementi di un solo quadro, che di fatto depotenzia gli strumenti cardine nella lotta alla criminalità organizzata. Insomma, in un momento storico come questo, in cui lo Stato ha il dovere di distribuire in modo oculato le risorse del PNRR, voi scegliete di indebolire la lotta contro le mafie e la corruzione. Severissimi con le persone più fragili: basti pensare alla fine del reddito di cittadinanza o alle norme abominevoli contenute nel decreto Caivano (il mancato rispetto dell'obbligo scolastico viene punito togliendo alle famiglie i quattro soldi del reddito di inclusione); molto più comprensivi, invece, con mafiosi e colletti bianchi corrotti. È una scelta decidere da che parte stare e la vostra mi sembra chiarissima. Come se non bastasse, sono state bocciate le proposte emendative per offrire maggiori risorse ai centri antiviolenza e alle case rifugio. Dite di voler contrastare la violenza maschile sulle donne, ma tutto quello che vi limitate a fare è inasprire le pene per chi commette il reato. Non stanziate un soldo, però, come nel disegno di legge Roccella attualmente in discussione alla Camera. Fingete di non capire quanto sia importante la prevenzione e la formazione degli operatori e investire in esse e quanto sia di fondamentale importanza sostenere, con risorse adeguate, i centri antiviolenza e le case rifugio, che sono il primo approdo a cui una donna si rivolge disperata, ricevendo sostegno legale e psicologico, e una vera alternativa alla violenza. Per questi motivi, chiamati ad esprimerci sulla fiducia al Governo, noi di Alleanza Verdi e Sinistra non possiamo che opporre un forte "no". Sono moltissime le motivazioni politiche che ci inducono a respingere la fiducia a questo Governo, dalle disumane scelte in tema di immigrazione al rifiuto di approvare il salario minimo per legge, che aiuterebbe milioni di lavoratori italiani, allo smantellamento della sanità pubblica, all'assenza di politiche sul diritto di abitare, all'inadeguatezza mostrata a tutta Europa sul PNRR, alle scelte sbagliatissime in tema di disagio giovanile. È un voto contrario forte e netto, tanto più che posto su un provvedimento come questo. Una decretazione d'urgenza su temi eterogenei e non urgenti, affrontati in modo che non condividiamo affatto nel merito e nel metodo.

da un assunto: la natura di un Governo e la natura della sua maggioranza, il loro atteggiamento, il loro loro contenuto e modo di essere, si interpretano non soltanto dalle cose che un Governo e una maggioranza fanno, ma anche da come essi cercano di raggiungere gli obiettivi che si sono dati. decreto-legge che andiamo a convertire con questo voto di fiducia è proprio un esempio preclaro delle modalità da questo Governo, che sono fondamentalmente irrispettose della natura parlamentare della nostra Repubblica. Posso dire, senza tema di essere smentito, che

il titolo del decreto-legge perché merita; esso reca disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero delle tossicodipendenze, di salute, di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. Basterebbe questo per capire che dell'articolo 77 dell'articolo 77 si è fatta carne da cannone - per così dire - perché se il provvedimento si occupa di tutta questa roba, evidentemente non era né necessario né urgente. Vuol dire che esso è stato considerato una sorta di veicolo *omnibus* nel quale infilare qualsiasi cosa ci fosse da fare in quel momento.

Io ricordo che nel 2019 la Corte costituzionale ha detto che ciascuno di noi ha il diritto di ricorrere con un conflitto di attribuzione nel caso in cui la nostra funzione legislativa non venga tutelata. E questo è il caso,

e questa è un'altra pessima abitudine di questo Governo, che io non mi stancherò di denunciare. La norma penale non si delibera, non si assume, non si adotta in forza di un decreto-legge - signora Presidente - non è ammissibile. Lo so che è tecnicamente possibile, che la Costituzione non lo esclude, ma è lo spirito della Costituzione che lo esclude, se non lo fa la lettera della Costituzione, perché la norma penale incide sulle libertà dei cittadini e necessita per sua natura e necessita per sua natura di riflessione, di ponderazione, di equilibrio, di ragionamento. Bisognerebbe svolgere delle audizioni, sentire gli esperti e invece qui si approvano continuamente norme penali in forza di decreti-legge. Abbiamo cominciato con i *rave party*, la più grande emergenza del Paese, e poi ne abbiamo visti altri come il decreto-legge Cutro. Questo

perché avete i manettari e avete i garantisti. Quindi, ci mandate in Aula il signor Ministro, le cui idee garantiste noi peraltro sosteniamo con grande entusiasmo, ma poi producete una figura di reato nuova al mese e aumentate le pene.

Decidete che anche per i reati di lieve entità si vada in galera se si tratta di sostanze stupefacenti, senza sapere, forse, che le nostre carceri esplodono. Fate un'analisi di impatto su che cosa significhino queste norme o pensate di risolvere tutto con nuovi reati e nuove pene? Ora dirò una cosa che probabilmente incuriosirà chi ci ascolta. In questo decreto c'è un nuovo reato,

già turbato dal ritirarsi dei ghiacciai e dal cambiamento climatico, ha anche delle norme della Repubblica italiana che lo discriminano rispetto all'orso marsicano.

di un'indagine conoscitiva sulle intercettazioni; abbiamo sentito decine di esperti, giuristi, tecnici, esperti informatici. Mentre il Senato fa tutto questo, alla Camera passa un decreto-legge che va in direzione contraria direzione contraria alle conclusioni dell'indagine conoscitiva, allargando le intercettazioni e per di più - e questo è gravissimo - in forma retroattiva, per decreto-legge. Io mi fermo qui, perché penso di aver detto tutto e di aver spiegato che atto di umiliazione sia questo modo di agire nei confronti del Parlamento. Penso altresì che qui si stia facendo strame, si stiano riducendo si stiano riducendo a nulla i principi delle garanzie costituzionali che sono scolpiti nella nostra bellissima Costituzione. È per questo - come dicevo - che non è sufficiente giudicare un Governo dalle cose che fa, ma da come le fa e questa volta, per come le ha fatte, noi voteremo contro la fiducia, con la massima convinzione e anche la massima preoccupazione, signora Presidente.

commessi con metodo mafioso. Era una richiesta che arrivava direttamente dalla Procura nazionale antimafia ed è stata accettata e fatta propria vogliamo aiutare i mafiosi o attenuare la lotta alla mafia viene frontalmente smentito da questa iniziativa dell'Esecutivo. Tuttavia, nel corso del dibattito alla Camera il testo è stato emendato soprattutto - riconosciamolo, colleghi - per merito di Forza Italia, che ha introdotto delle modifiche normative in tema soprattutto di intercettazioni. È stato ricordato da parecchi degli oratori che mi hanno preceduto il grandissimo lavoro che è stato svolto qui al Senato in Commissione giustizia, sotto la guida sapiente della presidente Bongiorno, in tema di intercettazioni. E mi è dispiaciuto che taluno dei colleghi intervenuto stamane qui in Aula e anche in Commissione abbia cercato di banalizzare quel lavoro con riferimento alla portata di questo decreto-legge, bollandolo come pura accademia o semplice convegno giuridico. In realtà, colleghi, il lavoro che è stato prodotto in quella indagine conoscitiva e le conclusioni che sono state approvate trovano riferimento proprio in questo testo. Mi riferisco in particolare alle modifiche introdotte in materia di intercettazioni a catena o a strascico. Su questo tema credo che i colleghi Bazoli e Scalfarotto debbano darmi atto che naturalmente è stata una conclusione condivisa quella di ritenere È proprio quello che è stato ottenuto alla Camera, con un dibattito

Con riferimento a queste intercettazioni si adotta un principio più restrittivo, che era quello riferito anche alla legge Orlando, interpretato dalla Corte di cassazione, anche in questo caso con un *caveat* riferito al fatto che questo tipo di interpretazione (sentenza Cavallo) non riguarda i reati più gravi, non quelli di mafia e terrorismo e, quindi, si applica quello che noi abbiamo tante volte chiamato il cosiddetto doppio binario. Ricordiamo - questo per dire come l'impostazione politica e giuridica sia completamente diversa - che, a fronte della sentenza Cavallo del 2 gennaio 2020,

si era subito attenuata una portata che - lo ripeto - nasceva dal combinato disposto della cosiddetta legge Orlando e della interpretazione delle sezioni unite della Suprema corte di cassazione. In questo senso, credo che si possa dire che il risultato condiviso della nostra indagine conoscitiva ha trovato trasposizione all'interno di questo testo di legge per iniziativa di un partito garantista qual è certamente Forza Italia. Mi è dispiaciuto qualche riferimento che è stato fatto poc'anzi nella discussione generale, con argomentazioni giuridiche non pertinenti, con riguardo al principio introdotto con un emendamento sempre alla Camera, ossia

anche a favore dell'indagato - e niente brogliacci per quanto riguarda le intercettazioni non rilevanti. Questo per evitare quella discrezionalità del maresciallo che possa in talune occasioni orientare le indagini o l'opinione pubblica. Proprio oggi, colleghi, leggendo le cronache giornalistiche, si ipotizza che sia stato un esponente delle Forze dell'ordine a diffondere le immagini *hot* del sindaco di Santa Marinella Tidei. Ciò per dire il pericolo che i brogliacci e le intercettazioni possano essere gestite dalla Le intercettazioni che non vengono trascritte nei brogliacci non vanno, però, perdute. Mi dispiace contraddire la collega Rossomando, che è sempre precisa studiosa, ma esse non vanno perdute, poiché rimangono nell'archivio segreto e gli avvocati e i periti potranno comunque consultarle, senza però passare attraverso quell'arbitrio costituito dalla valutazione del tutto discrezionale della polizia giudiziaria per quanto riguarda la trascrizione dei brogliacci. Altro principio che è stato applicato ed è contenuto in questo decreto-legge, a seguito di un emendamento di Forza Italia, è quella motivazione rafforzata che viene oggi richiesta per i captatori informatici, ossia il famigerato *trojan*. Di esso ci siamo molto occupati in sede di indagine conoscitiva. Tutti gli esperti ci hanno detto che è un prodotto assolutamente delicato, in continua evoluzione, che si presta anche a delle manipolazioni. Da qui la nostra cautela, che abbiamo espresso in diverse occasioni, per l'utilizzo di questo meccanismo di indagine così intrusivo. Nel corso del dibattito alla Camera, o meglio a margine del dibattito alla Camera, il ministro Nordio ha annunciato un intervento prossimo da parte del Governo di riordino della materia. E di questo ci compiacciamo perché - come qualcuno ha ricordato - nell'indagine conoscitiva conoscitiva presso la Commissione giustizia proprio Forza Italia ha richiesto che fosse inserita tra le conclusioni una richiesta di approfondimento e riflessione, anche alla luce non di arbitrarie argomentazioni, ma di una recentissima ma illuminante sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 7 settembre scorso. Tale sentenza ha stabilito un principio che noi reputiamo assolutamente

mentre per l'utilizzo del *trojan* è necessaria una motivazione rafforzata. Credo che questo sia un elemento di assoluta garanzia per il cittadino, che va nello spirito delle conclusioni di quella indagine conoscitiva che abbiamo svolto in Commissione giustizia. Quindi, signor Presidente, certamente Forza Italia voterà la fiducia al Governo e voterà a favore di questo decreto-legge, perché al suo interno si possono cogliere quei principi di garantismo giuridico che fanno parte del nostro DNA e per i quali ci battiamo costantemente.

Più va avanti la mia nuova esperienza di senatore, più sono costretto a prendere atto di quanto si vadano progressivamente svuotando il ruolo e la funzione dei parlamentari e sempre più mi sembra di essere una sorta di figurante di una democrazia recitativa, cioè svuotata di reale sostanza e ridotta a un mero rituale recitativo messo in scena per il pubblico. Il dibattito di oggi sul disegno di legge di conversione è paradigmatico di questo processo di progressiva erosione della democrazia parlamentare, come prevista dalla nostra Costituzione, e della sua surrettizia sostituzione con una nuova Costituzione materiale, che procede a tappe forzate e senza validi anticorpi nella direzione della marginalizzazione del Parlamento e della crescita anomala e ipertrofica dei poteri del Governo. Il disegno di legge è stato incardinato ieri alle ore 14; sono state concesse ai senatori solo due ore e mezzo, sino alle ore 17,30, per lo studio e la presentazione di emendamenti; sicché personalmente alle 17,30 sono rimasto con la penna in mano perché era scaduto il termine per scrivere gli emendamenti. Sappiamo tutti che il dibattito di oggi, ove pure si fosse svolto sui singoli emendamenti, sarebbe stato puramente formale, perché non ci sarebbero stati i tempi per un reale e produttivo confronto, e che la scelta di porre il voto di sfiducia si limita a stracciare ogni velo di ipocrisia e a rendere pubblico che il Senato è ridotto a luogo di ratifica notarile di decisioni già prese altrove. Mi permetto di dubitare che tutti i senatori presenti abbiano un'esatta cognizione delle norme che si apprestano a ratificare per disciplina di partito. Quanti - per formulare un solo esempio - si rendono conto che si sta approvando una norma che scrimina penalmente attività illegali delle Forze di polizia, consistenti nell'introdursi all'interno di un sistema informatico telematico, danneggiandolo, alterandolo, attivando false identità digitali, assumendo il controllo occulto dello spazio informatico dei cittadini? Quanti lo sanno qui dentro? Com'è possibile ritenere che si possa approvare a scatola chiusa una norma che attribuisce poteri così incisivi e gravidi di conseguenze sui diritti dei cittadini senza che vi siano stati il tempo il modo di discutere e meditare emendamenti che garantiscano e documentino una piena tracciabilità *a posteriori* degli interventi manipolativi e informatici effettuati? Quanti si rendono conto che stanno approvando con lo strumento della conversione di un decreto-legge una norma sulla salvaguardia degli orsi marsicani, qualificando questo intervento legislativo come un caso straordinario di necessità e urgenza ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione? *(Applausi)*. Vi sembra un modo serio questo di fare i legislatori? Non avrei fatto questa premessa se si trattasse di un caso sporadico o eccezionale, ma si tratta invece di un paradigma costante. Com'è già stato osservato da autorevoli costituzionalisti, dal momento in cui si è insediato, il Governo Meloni ha deliberato in undici mesi ben 39 decreti-legge, battendo tutti i *record* dei precedenti Governi per produzione mensile. La produzione legislativa di iniziativa parlamentare è quantitativamente e qualitativamente residuale; i decreti-legge vengono utilizzati come un ordinario strumento di produzione legislativa, come se si trattasse di disegni di legge, tant'è che ormai è prassi che il Governo preannunci di riservarsi di presentare emendamenti. È un vero e proprio esproprio della funzione parlamentare, tanto più se si tiene conto che nella maggior parte dei casi si tratta di decreti-legge *omnibus*, che riguardano le più svariate materie, e non sono affatto configurabili i casi straordinari di necessità e urgenza che, ai sensi dell'articolo 77 della Costruzione, legittimano l'adozione dei decreti-legge. esproprio della funzione parlamentare - spiace dirlo - avviene con la quiescenza passiva dei Presidenti della Camera e del Senato, che hanno abdicato alla loro funzione di garanti del ruolo della dignità delle Camere, trasformandosi in cinghia di trasmissione delle decisioni del Governo *(Applausi)*; abdicazione, questa, fortemente agevolata dal fatto che l'attuale maggioranza ha riservato a se stessa la Presidenza delle due Camere, rompendo la precedente pluriennale prassi che prevedeva che una delle due fosse assegnata alla minoranza. un esproprio della funzione e della dignità parlamentari che si realizza anche con la connivenza adesiva della maggioranza che sostiene questo Governo, divenuta complice dell'Esecutivo nel disegno di utilizzare decreti-legge come strumento ordinario di produzione legislativa, strozzando così i tempi e i modi del dibattito parlamentare e comprimendo oltre misura lo spazio politico delle minoranze. Si è dato vita a un perfetto gioco di squadra tra Governo e maggioranza governativa, che può essere sintetizzato nei seguenti termini: il Governo emana decreti-legge a getto continuo sui temi più eterogenei, dettando al Parlamento l'agenda dei lavori, e apre così corsie temporali di urgenza di appena sessanta giorni per la conversione in legge; le maggioranze parlamentari, a loro volta, approfittano di questa limitazione dei tempi e della compressione del dibattito parlamentare per salire sul carro in corsa ed effettuare veri e propri colpi di mano, inserendo nella forma mascherata di semplici emendamenti - e talora all'ultimo momento - nuove norme innovative e di grande valenza e impatto politico, sottraendosi così in modo sleale a un reale confronto sia nel Parlamento sia nel Paese. Esemplare è il disegno di legge di conversione di oggi: com'è noto, in Commissione giustizia al Senato è stata svolta un'ampia indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni, durata vari mesi, nel corso della quale sono state audite decine di esperti e che si è conclusa con una relazione nella quale si è dato atto di vari profili problematici, proponendo soluzioni aperte, che avrebbero poi dovuto essere discusse in un successivo dibattito parlamentare. Tutto tempo sprecato e carta straccia: avremmo potuto risparmiarci la fatica, con un colpo di mano, poco prima della scadenza dei termini di conversione in legge di questo decreto-legge, alle Camere le forze di maggioranza hanno introdotto modifiche rilevantissime agli articoli 267, 268 e 278 del codice di procedura penale sulle intercettazioni, sottraendosi così a un serio confronto non solo in Parlamento, ma anche nel Paese. *(Applausi)*. Ed è proprio grazie a questo sleale colpo di mano, all'abuso della forza dei numeri e allo svilimento del Senato che entreranno così in vigore norme che costituiscono gravi violazioni dei diritti dei difensori degli indagati e che allargano ulteriormente gli spazi di impunità per i reati dei colletti bianchi. È stato introdotto il divieto di trascrivere anche sommariamente il contenuto delle conversazioni intercettate ritenute non rilevanti per le indagini. E, poiché nessun pubblico ministero ha il tempo di ascoltare personalmente ore di intercettazioni è stato così attribuito al personale di polizia addetto all'ascolto - si alterna e a volte non conosce neanche le linee portanti delle indagini - il compito delicatissimo di stabilire quali conversazioni siano rilevanti per l'accusa e quali per la difesa. E ciò avviene senza che vi sia la possibilità di consentire *a posteriori*, sia al pubblico ministero sia agli avvocati, di verificare se sia stata omessa la trascrizione sintetica di contenuti intercettivi rilevanti per l'accusa e la difesa, perché delle conversazioni che la polizia ha ritenuto di qualificare non rilevanti non resta alcuna traccia e gli avvocati non si possono orientare. È stata introdotta una modifica dell'articolo 270, che consente l'utilizzazione di intercettazioni in altri procedimenti se si tratta di reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza, tipo i reati di strada come i furti aggravati, ma non consente l'utilizzazione di intercettazioni per i reati dei colletti bianchi, neanche quando vi sia la connessione probatoria, facendo un passo indietro rispetto alle sezioni unite della della sentenza Cavallo. Ecco, dunque, che questo non è un normale passaggio parlamentare. Questa è una tappa significativa, perché si è superato il limite della decenza istituzionale, sarà ricordata come un ulteriore scivolamento verso la degenerazione di questa democrazia e lo svuotamento della Costituzione. E siccome il MoVimento 5 Stelle è il partito che più ha a cuore la democrazia costituzionale, noi non ci stiamo e non votiamo questo decreto. ha facoltà. STEFANI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, questo disegno di legge di conversione del decreto-legge si inserisce nelle importanti tappe che anche il ministro Nordio sta portando avanti per una riforma della giustizia. Di certo non sono ignote al Governo, come si vede, infatti, proprio dalla formulazione stessa dei testi, le considerazioni che sono state svolte e anche le criticità che sono emerse, evidenziate nel corso dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni che è stata svolta in Commissione giustizia. Ringrazio la presidente Bongiorno, per l'efficienza e per come ha condotto sapientemente i lavori della Commissione, e anche tutti i membri della Commissione: quarantasette audizioni corpose, importanti, con auditi che vanno dal mondo

La relazione che è stata predisposta e approvata in Commissione ha dato infatti conto della necessità di un contemperamento degli interessi; interessi che sono le esigenze investigative, ma anche il diritto alla difesa e il diritto stesso all'informazione. Si è giunti, così, a una elaborazione che dovrà essere un riferimento per tutte le norme che dovranno essere approvate sul tema delle intercettazioni.

nonostante gli anni passati a parlare del tema delle intercettazioni. Intanto, sono stati riconosciuti degli strumenti anche più incisivi per la lotta contro il traffico illecito di rifiuti, il sequestro di persona, il terrorismo, prevedendo che vi siano limiti meno stringenti per le stesse intercettazioni, per poter quindi indagare e recuperare i mezzi della prova di reati. Poi, è stato affrontato un tema particolarmente delicato, che è l'uso del captatore informatico. Qualsiasi cosa si dica in merito, anche negli interventi che sono stati svolti, anche dalle opposizioni, noi ricordiamo che, fino a prova contraria, noi abbiamo una Costituzione, ma non solo quella, perché vi è anche la Corte europea dei diritti dell'uomo.

fortemente invasivi. Abbiamo avuto la prova e la dimostrazione, durante le audizioni, che certi *virus* - il *trojan* è sostanzialmente un *virus* inoculato - possono addirittura modificare i dati stessi contenuti all'interno dello *smartphone* o del *computer*. Quindi, potenzialmente, è uno strumento che ha addirittura questa capacità. La configurazione e la natura stessa del captatore informatico vanno oltre il tradizionale modo di pensare l'intercettazione (la classica intercettazione fra presenti, magari con la

nel disegno di legge è stato approvato un emendamento che prevede una motivazione rafforzata per l'utilizzo del *trojan*: occorre un'autonoma valutazione delle specifiche ragioni che rendono necessario, in concreto, lo svolgimento di un'indagine attraverso questa modalità.

Guardiamo anche a casi recenti, come i dialoghi di Zaia su Crisanti; cosa è stato scritto, cosa non è stato scritto, tutto buttato in realtà in un agone, per poi sfumare nel nulla. È un tema spinoso e difficile quello della divulgazione. divulgazione. A quale interesse obbedisce? È una vera necessità? È un vero diritto? O è soltanto un seguire, un ossequiare una pruriginosa curiosità collettiva del pubblico? Correttamente e doverosamente si è giunti quindi ad adottare questo tipo di provvedimento, che prevede che la trascrizione dei verbali sia limitata al contenuto delle intercettazioni rilevanti, evitando che vi siano delle

che già aveva stabilito un limite all'uso delle intercettazioni nei procedimenti diversi. Anche qui si è giunti a un ritorno, considerando la possibilità di utilizzarle solo quando sono indispensabili e quando ineriscono a delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

di legge è prevista un'aggravante per colui che commette l'atto con abuso di potere e con la violazione dei doveri. Perché scrivere questo? Signori, significa che c'è qualcuno che questo ha fatto.

Signori, noi non possiamo che confermare il nostro appoggio al Governo quando rivolge la propria azione, soprattutto in tema di giustizia, verso una riforma che necessita di coraggio, e non solo. Le vere riforme della giustizia non avvengono a costo zero e soprattutto non avvengono solo attraverso la continua e accanita tendenza a modificare inutilmente il rito. Abbiamo di fronte oggi l'entrata in vigore della riforma Cartabia, che è agli inizi e sta già evidenziando delle problematicità, che spero e auspico il Governo vorrà affrontare,

richiede e pretende un'analisi di un sistema e non solo degli interventi puntuali. Occorre concretamente ristabilire la vera indipendenza dei poteri, dove la funzione della magistratura è e dovrà diventare sacra, non solo per legge, senza dare adito a dubbi di influenze ideologiche come avvenuto anche recentemente su alcuni fatti. Non devono esserci nemmeno dubbi che vi possano essere delle decisioni ispirate a delle convinzioni ideologiche e politiche. In questa riforma la politica dovrà essere nobile e dovrà essere rispettata, ma per esserlo, dovrà prima di tutto rispettare. Colleghi,

poco gloriosa, anzi, se posso dire, umiliante per il Senato, per le nostre istituzioni e - se posso permettermi - per la nostra democrazia.

per trasformarci in impiegati ed esecutori della volontà del Governo senza alcun confronto, alcuna riflessione, alcun dibattito, alcun approfondimento.

Questo decreto-legge è stato approvato dal Governo l'8 agosto scorso ed è arrivato in Commissione ieri alle 14, quando è stato incardinato; esattamente ventiquattro ore fa. Dopo una breve illustrazione in Commissione, sono state date tre ore per depositare gli emendamenti. Tre ore per studiare, analizzare, verificare e lavorare sugli emendamenti.

Fine del nostro lavoro su questo decreto-legge. Una vera umiliazione per questa Camera, per il nostro Senato, alla quale io credo occorre che tutti noi, maggioranza e opposizione, ci ribelliamo. Non possiamo essere disponibili ad assuefarci a questo modo di lavorare. Nessuno nega alla maggioranza il diritto di governare, di far valere i propri numeri, di attuare il proprio programma, ma noi pretendiamo di essere messi in condizione di esercitare il nostro ruolo di opposizione, che è essenziale in una democrazia al pari di quello della maggioranza. Un ruolo nel quale ci troviamo oggi noi e domani potreste trovarvi voi in un'alternanza fisiologica in una democrazia. È infatti il ruolo di chi controlla, di chi discute, di chi si confronta nell'interesse di quella parte del Paese che rappresenta e che non è al momento maggioranza protempore. Tutto questo ci è stato negato. Ci è stato negato ieri, ci è stato negato oggi e noi pensiamo che questo uso smodato della decretazione d'urgenza

Non solo si sono compressi i tempi in misura tale da negare la nostra funzione, ma si è portato all'approvazione dell'Assemblea un provvedimento

di straordinarietà e di urgenza, cioè di tutti quei principi e quei criteri che sono stati posti dalla Costituzione e che poi sono stati anche sanciti dalla Corte costituzionale in numerose sentenze.

C'è tutto, è il decreto "la qualunque", dov'è l'omogeneità dei temi? Dov'è l'omogeneità delle questioni che dovrebbero essere inserite in un decreto? Sotto il profilo dell'urgenza, poi, è perfino peggio, perché voglio dire con chiarezza che è ora di smettere di usare la decretazione d'urgenza per intervenire sul diritto penale, sul tema più delicato che riguarda i diritti e le garanzie nel nostro Paese, è ora di finirla. Il decreto *rave*, poi il decreto Cutro, poi questo decreto, il decreto "la qualunque", tra poco il decreto Caivano sono tutti i decreti-legge con i quali si affrontano i più vari problemi, sull'onda di un'emozione o di un'emergenza e all'insegna di un'unica soluzione: aumentare le pene. Di fronte a qualunque emergenza, cioè, vera o supposta che sia, la soluzione è sempre la stessa: un bel decreto che inasprisce le pene, quando qualunque giurista sa bene e se non lo sa, è bene che studi o legga qualche tonnellata di ricerche in proposito o magari guardi la straordinaria efficacia del decreto Cutro, quello che ha aumentato le pene per gli scafisti e dopo il quale gli sbarchi sono triplicati

I fenomeni sociali devianti vanno affrontati in modo assai più articolato e complesso che non facendo leva sul diritto penale. Perché questo ostinato modo di legiferare? Lo ha spiegato assai bene l'attuale Ministro della giustizia, come ricordava stamattina la collega Rossomando, quando nell'intervista al «Foglio» di poche settimane fa ha candidamente ammesso che alzare le pene non serve a nulla se non a fare la faccia feroce per mandare un segnale all'opinione pubblica. Signori, questa è la più perfetta definizione del più deteriore populismo penale alla faccia delle garanzie del diritto penale minimo, dell'ipocrisia garantista continuamente evocata. Siete i nuovi campioni del populismo penale, che applicate a ogni fenomeno, salvo in un particolare settore del diritto penale, nel quale diventate i campioni del diritto penale minimo, anzi oserei dire microscopico, ossia i reati contro la pubblica amministrazione. È curioso, vero? E ancora, questo decreto interviene su una materia come le intercettazioni, sulla quale questo ramo del Parlamento - è stato detto da tanti - ha svolto un'indagine conoscitiva che è durata sei mesi. un'indagine accurata, complessa, nella quale abbiamo ascoltato decine di esperti e che ha portato a una relazione finale per molti aspetti condivisa, anche se piegata con un *blitz* finale in Commissione a un uso strumentale politico contrastante con i suoi risultati. Ora mi chiedo a cosa sia servita quell'indagine, quanto tempo abbiamo dedicato a un approfondimento evidentemente inutile, se poi anche quel tema così delicato e importante viene viene affrontato con la mannaia del Governo, con la decretazione d'urgenza, con emendamenti inseriti all'ultimo minuto e poi approvati con la fiducia. Non è anche questa un'umiliazione del nostro lavoro, della nostra Commissione, della nostra funzione? Presidente, noi voteremo contro questo decreto. Ci ribelliamo e ci ribelleremo sempre a questo metodo che ci impedisce di svolgere il nostro lavoro e rimarremo sempre - noi sì - un vero e saldo presidio a tutela delle istituzioni, della democrazia, delle garanzie e dei diritti del nostro Paese. Signora Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, ormai non mi meraviglio più di niente, non vi nascondo che non mi illudo più, però non ho perso la speranza

però quando è costruttiva probabilmente può essere anche utile alla causa; quando invece è puramente strumentale, purtroppo, non serve assolutamente a niente.

che abbiamo approvato, come ricordava prima il collega Berrino, è stato proprio il cosiddetto decreto-legge *rave*, con cui non volevamo bandire la musica, non volevamo dire no alla musica; volevamo cercare di disciplinare l'organizzazione della musica e principalmente volevamo trasmettere un messaggio a voi per farvi capire che la musica è cambiata, cari signori, e dovreste cercare di farvene una ragione. Perché si continua a parlare di urgenza? Molto probabilmente abbiamo un concetto diverso di urgenza. Voi la paragonate solo alla fretta, noi invece la

Egli infatti ha detto: dopo quello che è successo dei miei amici mi hanno consigliato anche di scrivere al Presidente del Consiglio, ma io ho scritto a tutti negli anni, addirittura al segretario del Papa, ma non ho mai avuto risposte. E poi lui stesso ha ammesso che dopo un mese sono arrivati a Caivano il Presidente del Consiglio, i Ministri, il Governo nella sua interezza, il Capo della Polizia e dopo qualche giorno le ruspe. Questo è il nostro modo di lavorare, con quell'operatività a risolvere i problemi, perché noi apparteniamo al Governo del fare. *(Applausi)*. La differenza è sostanziale e proprio perché apparteniamo al Governo del fare, vogliamo fare e lo facciamo con una certa urgenza. oggi è quello delle intercettazioni. Nei mesi scorsi siamo stati accusati, o meglio il Governo è stato accusato di voler eliminare le intercettazioni: era una bufala che voleva favorire le mafie. Oggi invece ci accusate perché le intercettazioni vengono estese.

per abolire l'isolamento previsto dal periodo Covid? Non possiamo continuare a tenere l'isolamento previsto.

l'amministratore a più livelli, è un mio *modus operandi*. Ci avete accusato di essere arrivati in fretta, perché è un decreto-legge approvato il 9 agosto alla Camera e che scade il 9 ottobre al Senato, ma che solo ieri è arrivato

preparato in Aula, senza aspettare il *time out* di ieri, quando è stato incardinato in Commissione. Ecco perché parlo di critiche strumentali. Mi sarebbe invece piaciuto confrontarmi sul merito delle questioni. In questi ultimi tempi e nel mese di agosto abbiamo assistito, purtroppo, a quello che è successo in Sicilia e in Sardegna. Addirittura, gente che era andata a passare lì le proprie vacanze è stata evacuata da strutture turistiche per via degli incendi. Mi sarei quindi aspettato nel merito cosa avreste fatto, cosa avreste voluto fare al posto nostro, cosa ci avreste proposto. Invece, assolutamente niente. Io parto dal commissario della Protezione civile, il quale distingue in due fasi l'attività di prevenzione degli incendi, parlando di repressione e di prevenzione. Oggi ci stiamo preoccupando della repressione. Voi pensate che a noi tutti l'aumento eventuale di un ulteriore anno di reclusione dia

attraverso il quale poi scattano i vincoli di inedificabilità, che potrebbe essere una causa degli incendi; così come scattano i vincoli dell'inibizione al pascolo, che potrebbe essere anch'essa una causa. Ci meravigliamo degli anni di pena che vengono previsti? Proviamo a immaginare che cosa comporta l'incendio di un bosco piuttosto che di una foresta. Oltre al danno che si fa, c'è un danno ambientale, un danno alla salute, un danno paesaggistico, un danno alla collettività. Si tratta di boschi all'interno dei quali sono presenti dei percorsi, dei sentieri per *mountain bike*, per *trekking*, che naturalmente vengono distrutti, e se noi mettessimo insieme tutti questi danni probabilmente la pena sarebbe insufficiente. aver parlato della repressione, parlare anche della prevenzione; sicuramente ne parleremo, così come abbiamo fatto quando abbiamo affrontato il problema dei torrenti per il dissesto idrogeologico. Anche perché gli incentivi sono quelli che provocano e procurano il dissesto idrogeologico. Periodicamente dovremo fare l'aggiornamento di un testo coordinato, attualmente vigente per quanto riguarda la prevenzione incendi, e lì faremo le dovute proposte con la speranza di cercare di migliorare. Mi permetto di proporre che quello che stiamo approvando oggi in tema di sanzioni venga ben pubblicizzato anche attraverso le televisioni. Infatti, dobbiamo inculcare il pericolo nel quale si incorre, le responsabilità e quindi le sanzioni. fare anche delle pubblicità attraverso manifesti murali, perché la gente in qualche modo deve essere terrorizzata. Così saremmo sicuri che, molto probabilmente, prima di fare un'azione del genere ci si pensi non una volta, ma forse due.

attraverso venti droni, è riuscito a ridurre del 50 per cento gli incendi rispetto al 2022; si sono triplicate le persone intercettate, che sono state denunciate ed anche arrestate. ed anche arrestate. Questo per dire che mi sarebbe piaciuto effettivamente ascoltare delle proposte su tutti questi provvedimenti fatti da noi. Proprio perché noi siamo a sostegno del Governo del fare, confermo la volontà del Gruppo Fratelli d'Italia a votare favorevolmente la fiducia al Governo.

n. 105, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia: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

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. estratto a sorte il nome della senatrice Bevilacqua).* Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Bevilacqua.

Signor Presidente, intervengo perché ricordo perfettamente il 4 ottobre del 2019: ero nel mio ufficio al Ministero dello sviluppo economico quando il maresciallo Coppola, il mio capo scorta, venne da me per dirmi che era accaduto qualcosa nella questura di Trieste.

Insieme a lui, Pierluigi Rotta, trentaquattro anni. Entrambi vennero strappati alle loro famiglie da un assassino che riuscì a impossessarsi di una delle pistole di ordinanza e fece fuoco sui due agenti di Polizia. Ricordo un video virale che li rappresentava in vita, mentre stavano prestando servizio nel turno notturno cantando «Figli delle stelle» e mandando un messaggio a tutti i cittadini per dire loro che stavano vegliando sulla nostra sicurezza. Due agenti di Polizia che stavano semplicemente facendo il loro lavoro e che hanno perso la vita troppo presto in un modo troppo atroce. Mi voglio stringere ancora oggi alle loro famiglie. Ricordo l'allora questore di Trieste, Giuseppe Petronzi, oggi questore di Milano, il supporto che ebbe da tutta la città e la vicinanza di tutto il nostro territorio, ma credo di tutto il Paese in quei momenti così difficili alla questura di Trieste. È un momento di ricordo per due persone che che soltanto perché stavano facendo il loro lavoro sono state barbaramente assassinate. Questa sera sarò a Velletri, luogo di residenza della famiglia di Matteo Demenego, per portare il mio saluto personale a quella famiglia distrutta in quel in quel tragico 4 ottobre del 2019. Credevo fosse giusto ricordarli anche in quest'Aula.

si stesse per avviare in Aula la commemorazione del Presidente Napolitano. Quando io ho fatto presente che c'era stato dato troppo poco tempo per valutare il parere che era posto in votazione e che comunque si era a ridosso di un momento particolare in Aula e mi sono girata per uscire - ahimè - il presidente della 9a Commissione, senatore De Carlo, ha seguito la mia uscita con un gestaccio e con un labiale più che eloquente, ma non ripeto quello che ha detto. Credo che ciò sia gravissimo e che possa configurare addirittura una violazione del codice di condotta dei senatori,

sia lesivo del prestigio del Senato il fatto che un Presidente di Commissione si permetta di rivolgersi in questo modo a una senatrice che protesta per la compressione delle proprie prerogative parlamentari. Non sono intervenuta ieri perché sono venuta a conoscenza solo *a posteriori* dei gestacci inqualificabili del presidente De Carlo e mi auguro che si voglia stigmatizzare questo comportamento, perché non è la prima volta che parlamentari di maggioranza, non essendo magari in grado con l'intelletto di replicare alle legittime rimostranze dell'opposizione, ricorrendo a gesti e versi più degni di una stalla che del consesso del Parlamento. Presidente,da giorni nelle città universitarie gli studenti fuori sede hanno ripreso la mobilitazione avviata a maggio. Stazionano accampati nelle tende, davanti agli ingressi dei dipartimenti di ateneo e chiedono risposte. È una protesta civile, non violenta; è la determinazione di una generazione che non vuole più stare sotto ricatto e denuncia, di fronte all'opinione pubblica, il torto di dover sottostare alla mancanza di strumenti per poter continuare a studiare, la mancanza di residenze universitarie e politiche abitative, i costi da usura, sproporzionati e insostenibili, per l'affitto di una stanza o di un posto letto, ingigantiti dalla crescita fuori controllo dell'inflazione, del caro vita. In quelle tende c'è un pezzo di società, un pezzo di popolo e di futuro del nostro Paese. Studiare oggi in Italia è diventato un lusso per C'è un muro, una barriera sociale che impedisce ai figli delle famiglie povere o impoverite dalla crisi di andare avanti, di coltivare il proprio talento e la propria volontà. Quelle tende che alcuni commentatori e alcuni politici irridono sono invece un pugno nello stomaco per la coscienza di tutti, perché simboleggiano la peggiore delle ingiustizie. Un Paese che non investe nelle nuove generazioni non ha futuro. L'articolo 34 della nostra Costituzione afferma: «i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi». Mai come nella società di oggi per realizzare il proprio progetto di vita è indispensabile poter studiare, eppure questo diritto è negato a migliaia di ragazze e di ragazzi. Questa è una gigantesca questione sociale e su questo noi continueremo a fare una battaglia politica e parlamentare; continueremo a chiedere fondi per una legge sul diritto allo studio e il *welfare* studentesco, fondi per costruire alloggi universitari pubblici e non solo privati

agli affitti studenteschi; regole per dire basta alla speculazione del mercato immobiliare e alle storture della pratica degli affitti turistici brevi, che oggi impedisce agli studenti e anche a tante famiglie normali di poter vivere, di poter avere una casa a prezzi accettabili. Signor Presidente, in questi giorni sono andato all'università «La Sapienza» a portare solidarietà agli studenti. Tra le tende c'era un cartello con su scritto: «diritto alla casa è diritto allo studio». È una grande verità, che ne racchiude un'altra: per chi parte svantaggiato, il diritto allo studio significa tutto; significa abbattere i muri di un destino che non deve essere già scritto. Per questo, per la politica e per il Paese, non c'è sfida più importante e più urgente di quei ragazzi, in quelle tende. *(Applausi)*.